Signor Presidente, colleghi, Silvius Magnago si è spento ieri mattina a Bolzano, lasciando in noi un grande e incolmabile vuoto. Come Capogruppo dei senatori della Südtiroler Volkspartei voglio qui ricordare Silvius Magnago - il padre dell'autonomia sudtirolese - che ha rappresentato la guida politica, spirituale e morale della nostra Provincia in uno dei periodi più difficili della sua storia, e soprattutto il simbolo di pacificazione e di dialogo. Nel suo percorso politico ha attraversato anni difficilissimi, ma ciò nonostante si è dimostrato uomo di grande equilibrio, privilegiando sempre la trattativa, la mediazione e il dialogo e mai lo scontro. A lui e alla sua opera non dobbiamo soltanto lo Statuto d'autonomia in quanto tale, ma soprattutto la pacifica convivenza in una terra di confine in cui vivono popolazioni diverse per lingua e cultura. Vorrei brevemente ripercorrere la biografia politica di Silvius Magnago per rileggere la storia stessa della nostra terra, fortemente segnata dalla sua inconfondibile impronta politica. Tornato dalla guerra, diviene nel 1946 capolista della Südtiroler Volkspartei alle comunali di Bolzano, dove - eletto con grande maggioranza di voti - ricopre la carica di vicesindaco. Nel 1948 viene eletto primo presidente del Consiglio provinciale. Dal 1957 al 1991, viene nominato segretario del partito della Südtiroler Volkspartei, avviando un vero e proprio processo di modernizzazione della politica sudtirolese. Nel 1960 assume l'incarico come *Landeshauptmann*, presidente della Giunta provinciale, che manterrà per ben 28 anni, divenendo così il più importante ed autorevole rappresentante della Südtiroler Volkspartei, nonché il vero e proprio simbolo dell'intero territorio sudtirolese. Nei primi anni Sessanta sono numerosi i suoi interventi mirati a revisionare ed ampliare il pacchetto di autonomia, che in seguito verrà migliorato con il secondo Statuto di autonomia varato insieme ad Aldo Moro nel 1972. Nelle trattative a Roma si fa conoscere ed apprezzare come uomo politico affidabile, di parola e di alto profilo. Ceduta la sua "eredità politica" a Luis Durnwalder, è stato dal 1991 *Obmann* onorario del nostro partito. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la scomparsa di Silvius Magnago, all'età di 96 anni, viene a mancare il più importante testimone di un'epoca difficile per la nostra terra. A lui va tutta la nostra gratitudine perché, grazie al suo impegno politico e alla sua capacità di mediazione e di dialogo, la nostra Provincia ha potuto vivere decenni di stabilità e di crescita. Per riprendere il pensiero del Capo dello Stato, quest'uomo si è battuto con grande lungimiranza per far sì che il principio di valorizzazione delle autonomie locali confluisse in quel pacchetto di misure di speciale autonomia di cui fu autore e principale garante. Tra mille difficoltà e in periodi delicatissimi della storia del Südtirol, Magnago ha saputo agire nell'interesse di tutti i cittadini, ottenendo un modello di autonomia a difesa di tutte le popolazioni presenti nella nostra terra, che non a caso viene preso ad esempio in tutto il mondo. Concludo, ringraziando a nome del mio partito, per tutti i messaggi di cordoglio che gli sono stati rivolti dalle massime autorità nazionali ed internazionali, nonché dai massimi esponenti politici che hanno conosciuto Magnago di persona. Cito qui il senatore a vita Giulio Andreotti, che ha condiviso con lui le tappe più significative a Roma: «Scompare con Silvius Magnago una figura di eccezionale valore politico e morale alla quale le future generazioni dovranno rifarsi per costruire un avvenire solido e di profonda validità». Signor Presidente, onorevoli colleghi, la politica rappresentava per Silvius Magnago l'arte di orientarsi al possibile la politica rappresentava per Silvius Magnago l'arte di orientarsi al possibile senza rincorrere l'impossibile. Per noi resta e resterà per sempre l'esempio di un uomo democratico fedele ai propri principi morali e sociali. Un grande uomo, un grande europeista, un grande sudtirolese.

Presidente, colleghi, se dovessimo fare un paragone potremmo dire che la storia di Silvius Magnago è stata la storia del Sudtirolo e di tutto l'Alto Adige. Nasce, infatti, nel 1914

Quegli anni e il ventennio successivo sono gli anni in cui, di fatto, si creano le grandi lacerazioni nel mondo altoatesino, composto da quei nuovi italiani di madrelingua tedesca. Dopo il secondo conflitto mondiale è Magnago, l'uomo più in vista del nuovo partito della Südtiroler Volkspartei, a lanciare quel «*l**os**

infatti ricopre il ruolo di segretario della Südtiroler Volkspartei ininterrottamente dal 1957 al 1991. È sempre lui che conduce, con grande capacità e intelligenza politica, il passaggio dal «*l**os** von Rom*» al «*los von Trient*», ossia da quell'inizio di secessione dall'Italia alla richiesta di una vasta autonomia entro i confini italiani; cosa che del resto otterrà con il secondo Statuto di autonomia, a cavallo degli anni 1971-1972. Magnago - potremmo dire - ha vinto la sua battaglia storica. Lascia, chiaramente, in tutti noi un grande sconforto, ma anche un esempio, politicamente parlando, per la tenacia, lo stile con cui ha condotto le sue battaglie, la correttezza, l'intelligenza politica dimostrata e l'alta moralità; doti, queste, che hanno contraddistinto tutta la sua vita. Ai colleghi della Südtiroler Volkspartei e alla popolazione di tutto il Sudtirolo va dunque il nostro più sincero cordoglio.

Negli anni del Dopoguerra le autonomie e le specificità territoriali hanno vissuto momenti molto difficili, problematici. Magnago è stato un grande *leader*, importante non solo per l'Alto Adige, ma per tutte le altre particolarità territoriali come quella valdostana. Uomo di pace, fermo nel rispetto delle proprie peculiarità e nel riconoscimento dei diritti di una popolazione particolare, ma anche molto aperto al dialogo e desideroso di appartenere all'Italia. Se si parla molto di federalismo oggi è proprio perché la storia dell'Italia ha avuto dei grandi *leader* come Silvius Magnago. Pertanto, ci

Signor Presidente, a nome del Gruppo del Partito Democratico, esprimo vivo cordoglio ai colleghi senatori della Südtiroler Volkspartei e, per loro tramite, al presidente della Provincia autonoma di Bolzano, e a tutte le concittadine e a tutti i concittadini sudtirolesi per la morte del dottor Silvius Magnago. La sua figura e la sua opera di politico e di amministratore appartengono ormai alla storia di quella nostra Regione di confine: egli è stato un protagonista assoluto, durante decenni del secolo scorso fondamentali per l'evoluzione istituzionale, politica, economica e sociale del Südtirol. Credo che alla sua memoria possiamo rivolgerci con meritati attenzione e rispetto, anche per l'alto impegno politico che caratterizzò l'agire del presidente Magnago nelle logiche internazionali, garantendo un progressivo equilibrio tra le istanze locali (alcune delle quali si esprimevano in modo estremistico, ma egli ne prese le distanze), l'integrazione del Südtirol nel sistema costituzionale italiano, il ruolo di garante esterno riconosciuto all'Austria. Fu artefice di quel difficile, talora aspro, ma qualificante percorso politico che sfociò nel riconoscimento, con il cosiddetto pacchetto del 1972, di una più ampia, speciale autonomia alla Provincia di Bolzano nel contesto della Regione già prevista dallo Statuto approvato nel 1948 al termine dei lavori dell'Assemblea costituente. In quel lungo percorso, che lo vide sempre in prima fila e che ebbe uno snodo fondamentale nel raduno di Castel Firmiano del 1957 con la sua nuova parola d'ordine (il «*los von Trient*», che sostituiva il «*los von Rom*» ereditato dalla negativa esperienza fascista), il presidente Magnago seppe esprimere - insieme - la sua durezza di capo carismatico e la sua pragmatica flessibilità di abile dirigente politico. Il tutto innestato su una personale moralità ed onestà che lo ha comunque fatto apprezzare da chi, pure, lo contrastava. In questo momento di dolore per la comunità sudtirolese credo doveroso esprimere partecipazione per la morte di un uomo che fu artefice dei positivi destini di una porzione importante e significativa della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in attenta, intelligente e costante interlocuzione con le istituzioni repubblicane.

all'interno di una Provincia, quella di Bolzano, e di una Regione, quella del Trentino-Alto Adige/Südtirol, non esito a definire statista.

Va detto che di questa Provincia e, in parte, di tutta la Regione ha saputo guidare i destini di un'intrigante collettività umana e politica. Ricordo che oggi il Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel suo complesso, conta poco meno di un milione di abitanti.

decisamente unica in Italia. Questa società mistilingue è cresciuta insieme grazie alle prerogative costituzionali attribuite dall'Italia e al riconoscimento dei principi autonomistici garantiti dall'Accordo di Parigi, prima, e poi sanciti anche dall'Unione europea. È cresciuta È cresciuta in pace grazie, almeno negli ultimissimi anni, soprattutto alla capacità di dialogo di uomini di buona volontà, tra i quali sicuramente, in primo piano, si può annoverare Silvius Magnago, nonostante il percorso non sia stato del tutto tranquillo e faremmo torto, credo, alla sua memoria se non ricordassimo, accanto ai progressi compiuti dalla sua azione di mediatore anche giorni decisamente drammatici.

purtroppo, anche carabinieri, poliziotti e alpini posti a difesa dell'integrità nazionale su quel difficile confine. Era l'opera di gruppi terroristici sanguinari, limitati, ma determinati, contro i quali Magnago seppe schierarsi con decisione e con coraggio, anche se non riuscì a contrastare fino in fondo il loro disegno di secessione, di liberazione totale, come dicevano, del Südtirol dalla sovranità dello Stato italiano; una situazione garantita, come dicevo, dall'accordo De Gasperi-Gruber, all'alba della nostra Costituzione. Lo sganciamento dell'Alto Adige/Südtirol dal Trentino e la creazione di due Province totalmente autonome, all'interno di una Regione ormai diventata un baluardo di cartapesta, è frutto è frutto di un impegno forse più politico che amministrativo ed ha finito per avallare indirettamente una spinta secessionistica che, purtroppo, ancora oggi trova qualche riverbero, anche se fortunatamente oggi non si verificano più casi di violenza, anche se c'è ancora chi soffia sulla brace sotto la cenere, come, ad esempio, la signora Eva Klotz, figlia del più sanguinario dei terroristi degli anni Sessanta, da molti anni

fino in fondo la spinta liberatrice del Südtirol dall'Italia. Quindi, un'incapacità totale di analisi politica, ma aggiungo anche un'assenza totale di pietà cristiana e di umanità in persone come queste. Un po' di corda, a dire la verità, Magnago l'aveva data ai terroristi in quel momento, quando, in un momento di scoramento, disse: "Credevano che non vi fossero alternative agli attentati e, diciamola tutta: un pizzico di ragione forse l'avevano". Ecco, questa frase era stata alimentata, in particolare, da quel simbolico

via dall'Italia, via da tutto! Creiamo una cosa unica solo per noi!". Magnago fortunatamente seppe riconvertire quel grido in parole di dialogo, in particolare, come è stato ricordato, con Giulio Andreotti e con rappresentanti politici locali, grazie ai quali riuscì a tessere quella rete di intese capaci di evitare una crisi più lunga e più grave. Come testimone di quegli anni difficili, ma anche dello straordinario sviluppo sociale ed economico di cui oggi gode

con il proprio ammonimento gli amministratori di quella Provincia, come a confermare che nei giorni dello scontro più duro, fu giusto, fu provvidenziale privilegiare la ragione sulle passioni dell'estremismo.

anche personalmente*,* ho avuto occasione di ricordarlocome un *leader* importante, impegnato a garantire l'autonomia dell'Alto Adige e la valorizzazione del multilinguismo e del pluralismo etnico, ma nel quadro dell'unità del nostro Paese e della costruzione di una comune Patria europea. Com'è stato detto, uomo del dialogo, del confronto e della trattativa, ha contribuito a costruire un modello di autonomia solo ha consentito di rafforzare la convivenza e la coesione nel nostro Paese, ma che - è vero - è guardato con attenzione anche all'estero. Questo è stato il contributo che resta nel patrimonio storico e politico, e non soltanto del nostro Paese. sono presenti in tribuna gli studenti della Scuola media «Salvo D'Acquisto» di San Salvo, in provincia di Chieti. A loro rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la vicina conclusione dell'anno scolastico.

una nuova emergenza relativa alla Regione Campania. Dagli atti risulta che vi siano oltre 600 demolizioni esecutive derivanti da sentenze passate in giudicato con tempi e modalità differenti, siano 60.000-65.000 i procedimenti in atto che porteranno a demolizioni.

Per verità e giustizia politica dobbiamo spiegare perché si è giunti a questa emergenza, perché cioè il Governo è dovuto intervenire. Lo dico, colleghi, perché non vorrei che qualcuno fosse tentato di giudicare questo provvedimento come se non fosse - come invece è

perfino da autorevoli esponenti della magistratura campana, che hanno auspicato un intervento statale per gestire una situazione che è giunta sul piano dell'emergenza di ordine pubblico. potremmo inquadrare il provvedimento in una logica di sussidiarietà, anche se purtroppo non di quella sussidiarietà nobile di cui si discute nei convegni e della quale è ricco il confronto politico, quel modello di sussidiarietà verticale o orizzontale su cui rifondare un nuovo patto istituzionale e un modo per essere più vicini alle esigenze dei cittadini. La sussidiarietà che questo Parlamento ha già conosciuto, proprio con la Regione Campania, è quella frutto dell'incapacità di una Regione che costringe lo Stato ad un intervento, perché questa non è stata in grado di sovraintendere alle proprie competenze. ai fatti, con decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, l'allora Governo della Repubblica ed il Parlamento approvarono un condono edilizio relativo ad immobili realizzati prima del 31 marzo 2003. Certo, il condono fu molto dibattuto e fu oggetto di scontro politico e istituzionale, che portò anche alcune Regioni ad impugnare il provvedimento dinanzi alla Corte costituzionale. Ricordo che la Corte si espresse sulla legittimità del condono stesso, in quanto collegato ad una riforma della materia edilizia che ne fondava e ne giustificava le ragioni. La legge sul condono prevedeva un termine entro il quale le Regioni potevano-dovevano legiferare per realizzare il pieno diritto di esprimersi di esprimersi in una materia di tipica competenza regionale come il governo del territorio, per cui vi era anche allora competenza concorrente. La Campania non fu tra le Regioni che impugnarono il condono; non fu, come spiegherò, tra le Regioni che diedero attuazione alle loro competenze, e questa è una delle principali ragioni della situazione di emergenza che oggi abbiamo dinnanzi. Dapprima la Regione Campania fece una delibera di Giunta regionale in cui, sulla base delle funzioni di indirizzo e di coordinamento relative alla pianificazione territoriale, decise che la legge dello Stato non si applicava sul con una delibera di Giunta regionale si escludeva l'applicazione di una legge dello Stato. Stante le competenze di coordinamento e di indirizzo della Regione nella pianificazione territoriale, della confusione che questa delibera di Giunta provocò, il Governo impugnò la delibera della Giunta regionale in cui si applicava il condono dinanzi alla Corte costituzionale, la quale, in data 24 giugno 2004, una decisione che è ricordata come la decisione più breve nel dispositivo della storia della Corte costituzionale. Gli autorevoli giuristi che sono presenti in quest'Aula sanno come la brevità di un dispositivo sia eloquente anche rispetto al modo *tranchant* con cui il giudice si esprime. La Corte costituzionale dichiarava che non spetta alla Regione Campania, attraverso una delibera di Giunta regionale, adottare un atto nel quale si nega efficacia, all'interno del proprio territorio, a un atto legislativo dello Stato. di questa prima decisione, che è del febbraio 2004 (ricordo che i termini per la presentazione del condono ai sensi della legge del 2003 andavano dall'11 novembre 2004 al 10 dicembre 2004),

con notevoli modificazioni, condizionava l'applicazione del condono sul proprio territorio e sostanzialmente ne impediva la realizzazione. La stessa Corte costituzionale, in relazione al ricorso presentato dalle altre Regioni (tra cui la la Toscana, l'Emilia-Romagna e l'Umbria), si era già espressa sul fatto che il termine che veniva affidato alle Regioni per legiferare era congruo e che, quindi, le Regioni

della sentenza della Corte costituzionale (che arrivò successivamente, negando la legittimità della legge della Regione Campania), commentava la mattina dopo la conferenza stampa della Giunta Bassolino: «C'è adesso da chiedersi che valore abbia una legge della Repubblica fuori dei termini previsti dalla Corte costituzionale fissati il 12 novembre». Ricordiamo, infatti, che la Corte costituzionale aveva imposto alle Regioni il termine temporale massimo del 12 novembre per legiferare autonomamente in tema di condono.

Questa situazione ha provocato il fatto che in Regione Campania il condono edilizio non abbia mai operato. La ragione della mancata operatività del condono edilizio in Regione Campania è una delle cause dell'attuale

come non sfugge ai colleghi che conoscono la materia, non tutti gli abusi oggi oggetto di demolizione da parte dell'autorità giudiziaria sarebbero stati sanabili, ma una gran parte degli abusi che potevano essere sanabili (che la Corte costituzionale aveva detto che dovevano essere sanabili, avendo dichiarato la medesima Corte che il condono era legittimo) non hanno operato Qualcuno, nel dibattito, molto ricco, di questi giorni, ha fatto delle considerazioni che, sotto il profilo politico, possono anche avere un fondamento, ma sotto il profilo giuridico credo siano un insulto non solo all'intelligenza ma anche al rapporto di correttezza che le istituzioni devono avere nei confronti dei cittadini. È vero infatti che se qualcuno, nonostante il fatto che la legge della Regione Campania aveva impedito il condono, avesse presentato nei termini previsti dalla legge nazionale, avendo poi la Corte costituzionale dichiarato *ex tunc* la nullità della legge campana, quelle domande avrebbero dovuto essere ammesse. Ricordo ai colleghi che il condono prevede un'autodenuncia, una richiesta di sanatoria; un'autodenuncia relativa a un fatto che è qualificato dalla legge come illecito penale e che proprio le normative sul condono, per un certo periodo, a fronte del pagamento di una certa cifra, non rendono illecito penale: anzi, si paga una vera e propria oblazione per sanare il procedimento. Quindi, immaginare che i cittadini campani, certamente degli abusivisti, avessero potuto e dovuto presentarsi comunque come autodenuncianti di fronte ai Comuni sulla base di una previsione, molto ragionevole, che la loro Regione adottava un provvedimento illegittimo, credo sia una cosa non sostenibile. La sentenza della Corte costituzionale è del 2006; dal 2006 a oggi sono passati quattro anni; dal condono 2004 a oggi ne sono passati sei. La situazione di emergenza, che oggi ha portato il Governo e porta il Parlamento ad un'azione di proroga delle demolizioni, è maturata ogni giorno: è maturata prima con gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, poi con le sentenze, poi con le sentenze passate in giudicato, poi con le ordinanze di demolizione, adesso con le ordinanze di demolizione eseguite in danno dai Comuni per inottemperanza rispetto agli atti prodotti dalla magistratura. In questi sei anni, la Regione Campania e le Province della Regione Campania, che hanno la titolarità di alcuni fondamentali poteri sul controllo del territorio e anche sull'edilizia residenziale pubblica e sulla normativa e sulla normativa di settore, non hanno fatto nulla, lasciando incancrenire giorno per giorno una situazione che aveva e avrà un esito certo e scontato a fronte di una mancanza di intervento da parte di quell'organo - la Regione

tutte le altre Regioni ottemperare ai loro doveri e ai loro obblighi. Questa emergenza così incancrenita è soltanto della Regione Campania, che ancora una volta ha ha deciso volontariamente di non adempiere alle proprie funzioni, ha rinunciato ai propri poteri. Oggi questo intervento di sussidiarietà per supplenza è un atto di necessità di fronte a un problema di ordine pubblico che ha all'origine una responsabilità politica, colleghi, e una responsabilità istituzionale, esattamente come quegli stessi atti invasivi della competenza regionale che il Parlamento ha conosciuto nel tema della gestione dei rifiuti, per le quali le competenze sono delle Regioni e le competenze delle Regioni, qualora esercitate, non provocano una necessità di intervento da parte dello Stato, che invade in questo caso le competenze regionali di fronte all'incapacità della Regione. Questa è sussidiarietà atipica, che è la sussidiarietà campana, e che ancora oggi noi dobbiamo esaminare ed esercitare. C'è però un fatto nuovo. Perdonatemi se la metto su una questione politica, ma qui il tema è politico, anche in considerazione del fatto che dall'opposizione non abbiamo avuto un contributo né un riconoscimento rispetto a questo problema di emergenza, che è frutto di una maggioranza e di una Giunta amica, della quale anche alcuni colleghi sono espressioni territoriali: addirittura qualche ex assessore della Regione Campania è qui presente in Parlamento.

abbiano la possibilità di fare ciò che appartiene alle loro dirette competenze, ciò che oggi ha bisogno di un tempo minimo perché venga esercitato. Questo, per cercare di voltare pagina per il futuro ed evitare che il Parlamento si occupi ancora in questo modo della Regione Campania, invadendo le sue competenze e dovendo intervenire a fronte della conclamata e - se volete - condannata ufficialmente, dal corpo elettorale, incapacità di gestione di quel territorio che ha caratterizzato la Giunta Bassolino e gli ultimi

intendo illustrare la questione pregiudiziale anticipando fin da ora che appongo la mia firma all'ordine del giorno G100 (testo 2), presentato a prima firma dal senatore De Luca. Devo dire che l'ordine del giorno, per alcuni aspetti,

riferisco alla carenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, segnatamente nell'interpretazione che è stata fornita dalla Corte costituzionale nella misura in cui si introducono norme che ben avrebbero potuto essere oggetto di previsione attraverso l'ordinario *iter* legislativo in quanto il decreto-legge in conversione è diretto ad intervenire su situazioni ormai consolidate e tutt'altro che imprevedibili. L'ordine del giorno, tra l'altro, indica anche la Il secondo punto che intendo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea è che il decreto-legge in discussione sospende sino al 31 giugno 2011

in esame in ogni caso realizzano una irragionevole ed ingiustificata violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto circoscrivono gli effetti della sospensione ai soli immobili siti nella regione Campania. Questa delimitazione *ratione loci* della sfera di applicazione delle norme appare difficilmente compatibile con i principi sia di eguaglianza che di ragionevolezza che discendono dall'articolo 3 della Costituzione, nella misura in cui si attribuiscono si attribuiscono determinati effetti penali ad una medesima situazione non già in ragione della sua intrinseca offensività rispetto al bene giuridico protetto, ma unicamente in ragione del *locus commissi delicti*. Risulta tra l'altro - come dicevo - impossibile stabilire se gli abusi edilizi siano stati realizzati prima o dopo il 31 marzo 2003, termine stabilito dalla legge che ha disciplinato l'ultimo condono. La soluzione prospettata si rivela ancor più preoccupante per l'incapacità di verificare il momento effettivo della realizzazione degli abusi stessi e la stessa destinazione dell'immobile a prima indipendentemente da tutti i vincoli che, violati attraverso gli abusi, hanno prodotto effetti devastanti nella regione Campania. Ciò comporta, senza alcun dubbio, una grave situazione di incertezza, oltre che di manifesta ingiustizia e disparità di trattamento, in special modo in una regione, quale la

L'indeterminatezza delle situazioni che il decreto-legge dovrebbe regolare è tale da rendere quest'ultimo sostanzialmente inapplicabile e finisce con il favorire eventuali abusi commessi proprio in connessione con fatti di criminalità organizzata o comunque orchestrati dalla stessa camorra. Appare del tutto pretestuoso l'argomento per cui la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2004 avrebbe reso impossibile in Campania la presentazione di domande per accedere al condono. Inoltre, credo vi sia un aspetto particolarmente preoccupante: la prevista sospensione delle attività di demolizione disposte dall'autorità giudiziaria, in esecuzione di sentenze penali, rappresenta una palese violazione del principio della separazione dei poteri, poiché priva di efficacia pronunce giurisdizionali passate in giudicato, determinando un'indebita interferenza nell'esercizio della giurisdizione, con il rischio di delegittimarne l'operato della magistratura e di destituire di fondamento i principi della certezza dei diritto e della pena, nonché l'efficacia delle Grazie, la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge che, con una sorta di delega in bianco all'autorità amministrativa, finisce per far dipendere l'esecuzione di una sentenza penale dalla mera valutazione dell'ufficio amministrativo. Questo è davvero lo stravolgimento di principi fondamentali del nostro ordinamento su cui si fonda la nostra democrazia. Per contenuto, finalità e presupposti il decreto-legge in esame rappresenta una tipica legge provvedimento, ossia un atto sostanzialmente amministrativo privo quindi di quei caratteri di generalità, astrattezza e innovatività tipici degli atti normativi. Peraltro, diversamente dall'atto amministrativo, la norma primaria, anche se rappresenta una legge provvedimento, preclude agli interessati la tutela giurisdizionale delle proprie posizioni soggettive, con evidente ulteriore violazione del principio di uguaglianza e di un diritto inviolabile, quale quello di difesa, costitutivo dello Stato di diritto. Inoltre, bisogna considerare che il vero e grave problema sociale a cui il decreto-legge in esame non riesce a dare risposta dovrebbe essere risolto prevedendo una soluzione abitativa *ad hoc* per le famiglie interessate. A questo A questo mi sembra risponda perfettamente l'ordine del giorno. Non è pensabile affidare di continuo a provvedimenti di carattere emergenziale la soluzione di rilevanti esigenze sociali; a tale proposito, occorrerebbe tenere almeno ben distinto il caso di coloro che si trovano in oggettive condizioni di emergenza abitativa da quello in cui sono, invece, realizzati fenomeni di speculazione edilizia.

Per dare una reale e concreta soluzione ai gravissimi problemi abitativi presenti nella regione Campania, occorrerebbe agire nell'ambito di una visione organica del problema, prevedendo soluzioni alternative strutturali e non continuando ad operare in un'ottica emergenziale, di fatto infrangendo i principi di legalità.

combattevamo la mafia in territorio di Sicilia, tra le cose che cominciammo a sequestrare furono le imprese dei mafiosi. In quel momento i sindacati si opposero dicendo che i lavoratori avrebbero perso il posto di lavoro. Ci sono voluti molti anni perché la cultura della legalità si affermasse e fosse sostenuta.

e ciò non è accettabile per una democrazia. Quindi, insisto fortemente perché questa pregiudiziale sia accolta e perché si deliberi ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2144.

signor Presidente. Prima di iniziare il mio intervento, dichiaro il mio sostanziale accordo sull'affermazione, fatta dal senatore Orsi nella sua relazione,

ma si interviene semplicemente su una serie di sentenze penali che dovrebbero essere eseguite. La norma che prevede che possa esserci un autonomo intervento del giudice penale in materia di abusi edilizi non c'entra assolutamente nulla con le sentenze della Corte costituzionale e con il condono del 2003. È una norma che si muove autonomamente e noi sosteniamo che con questo decreto si vuole intervenire, ancora una volta, su delle sentenze che dovrebbero avere esecuzione, già pronunciate dai giudici legittimamente preposti a questo. È ben vero che esiste una differenza sostanziale tra il Governo attuale della Regione Campania e il Governo precedente. Non è un caso se il Gruppo del Partito Democratico non votò la la conversione del decreto n. 269 del 2003, che prevedeva il condono; non è un caso se la Giunta che ha preceduto questa ha ritenuto di dare un'impostazione restrittiva ai termini del condono nazionale. Ora, dal punto di vista dell'interpretazione giuridica è chiaramente giusto quanto ha scritto la Corte costituzionale, e io non interverrò su questa materia. Però, siccome il senatore Orsi ha detto che il problema è politico, si fronteggiano le due posizioni di chi immagina che i condoni edilizi possano avere una diffusione più ampia possibile sul territorio e di chi ritiene che, invece, si debbano restringere le possibilità di questo condono.

che esso nasce, apparentemente, per superare uno scontro di competenze legislative fra Stato e Regioni ma, in realtà, a quello non risponde. sa benissimo (e gliel'ho già detto in Commissione) che forse, per rispondere a quelle sentenze e a quelle esigenze, si doveva scrivere un altro testo di decreto (su cui io non sarei stata comunque d'accordo, perché non ero d'accordo sul condono edilizio iniziale). Non si può, però, pensare di intervenire su un pezzo, immaginando così di rispondere a tutti i problemi sollevati dalle sentenze della Corte costituzionale. D'altro canto, c'è ancora un altro problema: noi non sappiamo neanche quale sia il numero degli immobili che saranno sottoposti a questa norma. La relazione illustrativa del decreto parla di 600 casi. Dichiarazioni pervenuteci, a cui ha fatto riferimento anche il senatore Orsi, di esponenti della magistratura operanti in Campania forniscono il dato di 30.000, forse addirittura 60.000 casi. Ora è chiaro che le due cifre non sono assolutamente compatibili e non sono neanche paragonabili. Sarebbe forse stato opportuno che il Governo ci avesse dato almeno l'esatta entità del fenomeno di cui stiamo trattando. Qualcuno, tra l'altro, ha suggerito l'idea che l'entità del fenomeno sia così consistente, nei termini indicati dalla magistratura, perché molti Comuni campani sarebbero sprovvisti di piani regolatori o di piani di governo del territorio e, pertanto, non vi sarebbero aree edificabili per consentire la risoluzione del problema abitativo. In realtà, bisognerebbe chiedersi perché ci siano intere aree del Paese, e purtroppo non solo in Campania, dove l'assenza di legalità si manifesta ad ogni livello, in modi vari e nei più svariati settori. Amministratori, infatti, che non governano il proprio territorio e che creano contesti in cui i comportamenti illegali dilagano sono uno degli aspetti di questo grave problema. Noi pensiamo sempre alla grande malavita organizzata, ma dobbiamo ricordare che questa malavita interviene su un tessuto favorevole. Bisogna offrire ai cittadini un di più di legalità, perché solo nella legalità i diritti, in questa fattispecie il diritto alla casa, dei cittadini possono essere esercitati con pienezza e nel rispetto della legge. Diciamo che forse i deliberati dell'allora Giunta regionale della Campania, anche se magari non saranno stati perfetti dal punto di vista giuridico, tuttavia andavano in questa direzione. La differenza notevole tra le varie Regioni italiane non va assunta solo come un acritico elogio del Nord e un'altrettanto acritica condanna del Sud, immaginando per il Sud una punizione continua, come pensano talune forze politiche, bensì dovremmo interrogarci sulla diminuzione, quando non cancellazione, dei diritti dei cittadini del Sud dentro un contesto ambientale segnato da profonde illegalità e da istituzioni inadeguate rispetto ai compiti che dovrebbero assolvere, istituzioni inadeguate perché inadeguati sono gli uomini che le occupano. occupano. Se si vuole giustificare l'alto numero di abusi con il fatto che non esistevano i piani regolatori o i piani di governo del territorio, bisogna fare un esame attento di quello quello che sono stati gli amministratori, di quello che le istituzioni non hanno dato ai cittadini, altrimenti cadiamo nell'eterno errore di dire che c'è un Sud sempre e comunque fuori da ogni regola e un Nord che, come dicevano i giornali in questi giorni, ha una minor propensione a disattendere le leggi dello Stato. Ancora, può una norma come questa sanare i problemi che abbiamo davanti? E ancora, un'ulteriore domanda: perché queste demolizioni sono state disposte solo dall'autorità giudiziaria? È vero, lo dicevo prima: c'è una parte della disciplina che permette l'autonomo intervento del giudice penale e tuttavia mi chiedo: perché gli organi amministrativi non hanno fatto la loro parte? parte? Sia chiaro che se gli organi amministrativi avessero fatto la loro parte, probabilmente l'intervento del giudice penale si sarebbe manifestato in un minor numero di casi, questo è fuori da ogni dubbio. E allora vogliamo affrontare la questione di quali uomini per quali istituzioni una volta per tutte, oppure no? È possibile che in alcune parti del Paese gli amministratori colpiscono subito irregolari comportamenti edilizi dei loro cittadini ed in altre parti non se ne curano, immagino per non nobili motivi d'interesse elettorale quando non per palese disprezzo delle leggi? Paradossalmente si crea una non condivisibile Costituzione materiale che sancisce una disparità di trattamento tra cittadini di Comuni dove l'illegalità dei comportamenti è perseguita anche in sede amministrativa e cittadini di Comuni dove questo non accade. È chiaro che non sono contraria al rispetto pieno della legge, anzi io voglio il rispetto pieno della legge e lo voglio in tutti i Comuni, ma la deriva di provvedimenti come questo in esame conduce appunto ad una specie di violazione continuata del principio costituzionale secondo cui tutti i cittadini dovrebbero essere uguali davanti alla legge. Questo decreto dice che non è così, che non è così, ma non per colpa dei cittadini, bensì per il tipo di intervento che ogni volta si vuole adottare per sanare situazioni che sono insanabili. Il tema dunque degli amministratori è centrale. Non dovremmo in quest'Aula del Senato occuparci anche di loro, colpendo i loro comportamenti omissivi e illegali? Questo è un problema importantissimo Stiamo qui a discutere di sospendere delle esecuzioni penali perché gli amministratori e gli uffici tecnici dei Comuni non hanno fatto il loro dovere: mi pare una cosa degna di una certa attenzione. Questi comportamenti omissivi e illegali si sono verificati ben prima ben prima della legge sul condono e ben prima di questo decreto, perché quando si è arrivati al condono e al decreto i comportamenti omissivi ed illegali si erano già verificati e forse in certa misura continuano tuttora. In aggiunta,

ci sia un retropensiero, e cioè che il comma 2, che apparentemente è restrittivo, sarà sospeso in un limbo perché non troverà applicazione. Se allora immaginiamo questo, diciamo che il comma 2 dell'articolo 1 di questo decreto non avrà applicazione o scarsissima applicazione, perché lo affidiamo a quegli stessi che prima non hanno verificato quello che dovevano verificare. verificare. Ancora, si motiva questa norma come sanatoria di un problema sociale. Ma davvero - come recita la relazione accompagnatoria - le demolizioni aggraverebbero il già pesante deficit abitativo? Ma il deficit e l'emergenza

di sospendere le esecuzioni per gli immobili destinati a «prima abitazione». Il concetto di prima abitazione giuridicamente non sta da nessuna parte: nelle norme

non regaliamo loro sempre dei condoni assurdi. Credo che di questo abbia bisogno il Sud e di questo i cittadini meridionali ci saranno grati.

segnalo anzitutto il palese contrasto tra i riferimenti offerti dalla relazione accompagnatoria e la cognizione di causa emersa già nel dibattito in 13a Commissione: tanto la relazione prova a circoscrivere a poche centinaia di casi la questione quanto il testo del decreto‑legge e l'interpretazione del medesimo, offerta sia dal Governo sia dal relatore, ne estende sostanzialmente in modo indefinito l'applicazione (e sempre senza tener conto degli emendamenti depositati). Sono 600, 20.000 o 60.000 i casi soggetti all'applicazione della norma in esame? Come non sottolineare l'incongruenza e l'indeterminatezza giuridica del termine "prima abitazione", di cui al comma 1 dell'articolo 1; come non sottolineare l'incertezza giuridica connessa alla interpretazione del termine "soggetti sforniti di altra abitazione" pure contenuto nel primo comma dell'articolo 1? Come non rilevare la ipocrisia delle previsioni contenute nel comma 2 del medesimo articolo, laddove gli effetti demolitori di edifici conseguenti a sentenze penali vengono ripristinati su pronuncia dell'Ufficio tecnico del Comune, ovvero della Protezione civile regionale in ragione dell'accertamento di pericolo per la pubblica o privata incolumità, ovvero della violazione di vincoli paesaggistici. In questo secondo caso, poi, realizzando un curioso - per non dire altro - avvitamento normativo in confronto con la previsione del comma precedente, che sospende l'esecutività delle demolizioni in oggetto proprio per consentire - tra l'altro tra l'altro - una «adeguata ed attuale ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica», palesemente non di competenza di analitica rivisitazione da parte di un ufficio tecnico comunale. In realtà, siamo messi di fronte ad un'ipotesi di riapertura dei termini del famigerato condono dell'anno 2003, con la scusante della confusa situazione - che ci ha voluto ricordare il signor relatore - determinatasi a suo tempo nella Regione Campania a seguito di una delibera della Giunta regionale dapprima, e di una legge regionale successivamente, entrambe cassate in tutto o in parte dalla Corte Costituzionale. Secondo un consolidato modello adottato dalla attuale maggioranza, quella che - ad una lettura del decreto-legge - era, appunto, una ipotesi diventa ora esplicita certezza a seguito della presentazione di un impegnativo emendamento che addirittura largheggia in termini di condono sul territorio campano. Dopo il federalismo demaniale, abbiamo ora occasione di cimentarci in una sorta di federalismo "condoniale", dal quale non ci attendiamo nulla di buono, perché la maggioranza intende assentire in Campania ciò che altrove nel Paese non è ammesso. Non ci facciamo trarre in inganno dalla emergenza abitativa, per risolvere la quale basterebbe si attivasse positivamente la Regione, sottraendo quindi i meno abbienti al palese sfruttamento criminale dì chi costruisce ovunque mettendo avanti la povera gente, sanando facilmente il costruito e poi affittandolo o rivendendolo a caro prezzo, lasciando inalterato il bisogno sociale. E che dire degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici: chi li ha autorizzati, chi li ha pagati? Federalismo dell'arrangiarsi, oltre i limiti della legalità. Per una palese esigenza di equità verso chi si comporta diversamente, nel rispetto delle normative urbanistiche e verso quegli enti pubblici territoriali che fanno il loro dovere, sia nel controllo sull'attività edilizia, sia nella programmazione di piani per l'edilizia pubblica popolare ed agevolata, il giudizio che esprimo su questo decreto-legge e sugli emendamenti ulteriormente peggiorativi è del tutto negativo.

Non mi voglio addentrare nelle eccezioni di costituzionalità di questo decreto-legge che stiamo per convertire, perché non ne avrei nemmeno le capacità, non sono padrone della materia.

perché chiamato in causa per le inefficienze e l'incapacità della classe dirigente. Per molti amministratori

Questo ci mette nell'impossibilità di fare uno strumento agile e veloce che sia al servizio della comunità. un episodio per tutti. Nel 1983 in un Comune di 40.000 abitanti a nord di Napoli si mette mano, dopo il piano di fabbricazione che affondava le sue radici nel 1970, 1970, al piano regolatore. Nel 1985 viene licenziato e vengono arrestati 15 consiglieri comunali, compreso il sindaco. Successivamente, dopo un po' di anni, vengono tutti assolti, ma nel frattempo la Provincia aveva commissariato il provvedimento nominando un commissario *ad acta*. Nel 1998, 13 anni dopo, il provvedimento veniva licenziato, ma il redattore del piano intese abolire tutte le zone C, le lottizzazioni convenzionate.

cui era stato mistificato il valore dell'azione messa in campo, ha costruito abusivamente. Oggi, in forza di questo provvedimento, che voi rinviate alla Regione nella speranza che, come diceva Orsi, cambiata la maggioranza si possa legiferare in modo da poter sanare il sanabile e non tutto,

nel frattempo, per sentenza, il loro terreno è stato rivalutato; adesso non possono più avvalersi di quello che la legge avrebbe già dovuto concedere loro nel 1985. Ovviamente, in quegli anni ci sono stati gli abusi.

è stato stabilito per sentenza - non poteva essere fatto. Per la verità, non ho mai fatto ricorso come ultima *ratio* all'abuso e ho intravisto nel decreto-legge

colpevolmente assenti per nostra inefficienza. Nella disamina degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati mi sono reso conto, ahimé, che è

Pertanto, annuncio che il mio Gruppo non parteciperà al voto, ritenendo il provvedimento, così come emendato, eccessivamente permissivo rispetto alle ragioni di tanti, il cui il ricorso all'abuso, seppur deprecabile, andava in qualche caso compreso. Voglio dire un'ultima cosa. È chiaro che dobbiamo riformare la classe dirigente, perché non possiamo correre il rischio che le comunità paghino uno scotto per avere una classe dirigente non all'altezza della situazione. *(PD)*. Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame, nel prescrivere la sospensione per un anno delle demolizioni disposte dell'autorità giudiziaria di immobili abusivi destinati a prima abitazione siti del territorio campano, riferisce tale decisione, secondo quanto testualmente è scritto nella relazione di accompagnamento, a circa 600 casi, che coinvolgono altrettante famiglie e aggravano sensibilmente il già pesante *deficit* abitativo regionale. Subito qui osservo che la carenza di alloggi in Campania, come altrove, andrebbe affrontata in una visione complessiva e organica, a partire dalle cause che determinano l'assenza di un vero mercato degli affitti. Aggiungo poi che i casi specifici di famiglie che vivono in immobili abusivi dei quali è stata disposta la demolizione vanno gestiti dalle autorità amministrative competenti e va da sé che queste dovranno apprestare transitoriamente, per casi di bisogno reale e urgente, soluzioni alternative. Sarebbe invece a mio giudizio un grave errore

di fatto infrangendo i principi della legalità. A me pare che qui si stia rinunciando al ruolo dello Stato, che, in talune circostanze, deve assumere iniziative coraggiose ed esemplari che rechino in sé anche una forte valenza, per così dire educativa: la responsabilità delle classi dirigenti locali matura e si afferma anche su queste indicazioni. La relazione già innanzi citata richiama anche una sentenza della Corte costituzionale del giugno 2004, con la quale fu annullata l'efficacia di una deliberazione della Giunta regionale della Campania, adottata nel settembre 2003, attraverso la quale si negava sul territorio regionale l'operatività del condono edilizio, conformemente ad un precedente atto deliberativo della stessa Giunta approvato nel settembre 2002. Devo dire che è notevolmente fantasiosa l'interpretazione che il collega relatore dà dei fatti, dopo averne meticolosamente curato la ricostruzione. Ma soprattutto è abbastanza ardito pensare che intanto vi è l'abusivismo in Campania in quanto per iniziativa della Regione non è stato applicato il condono. È vero, semmai, un altro fatto: il proliferare di abusi edilizi dopo il 2003, nel tentativo di avvalersi del condono, questo sì. Ed è del resto scoperto il tentativo con cui, attraverso un emendamento, si vorrebbero riaprire i termini del condono 2003. Può essere condivisibile o meno da parte del relatore o di chi altri, fondato o no sul piano della costituzionalità relativamente prima alla competenza, poi allo allo strumento che la Regione utilizzò all'epoca per dissentire dal condono, ed ancora con riguardo alla cronologia degli eventi, meglio direi alla loro tempistica; sta di fatto però che il gesto della Regione fu innanzi tutto carico di significato e di responsabilità politici. Certamente, quel gesto fu impopolare negli esiti e assolutamente non remunerativo sul piano del consenso. Motivazioni queste ben evidenti e note alla maggioranza parlamentare di oggi, che le applica alla rovescia: infatti, essa sa bene quanto sia, viceversa, elettoralisticamente remunerativo il tipo di provvedimento oggi all'esame dell'Aula, che non per caso è stato oggetto di una premessa in epoca elettorale, durante la campagna per le regionali 2010. Se almeno si evitassero espressioni denigratorie verso l'istituzione regionale campana e chi l'ha retta sino a ieri, nonché all'indirizzo di una terra e di comunità ricche di storia, di tradizioni e di cultura come la Campania e come i campani, sarebbe già tanto! Al di là della sua fondatezza sul piano costituzionale, più che altro relativa - come ho detto - alla competenza in materia del soggetto decisore, la posizione assunta dalla Regione aveva anche un senso in rapporto all'elevata valenza ambientale del territorio,

nonché un territorio in cui sono presenti aree ad elevatissimo rischio vulcanico, sismico e idrogeologico e che dunque, per tutte queste buone ragioni e per le sue tante criticità, non può consentirsi distrazioni, non può avallare manomissioni. Basti pensare alla tragedia dell'alluvione di Sarno, di Siano, di Bracigliano, di Quindici e di San Felice a Cancello, il 5 maggio 1998 più recentemente, ai danni e alle vittime causate dal maltempo a Ischia e al distacco del costone roccioso di Atrani ad inizio anno, nonché al pericolo sempre incombente costituito dal Vesuvio ed aggravato dalla miriade di costruzioni alle sue falde, per rendersi conto di quale devastazione siano state capaci di produrre nei decenni passati, e nell'epoca più recente, una dissennata gestione del territorio - lo dico con chiarezza e me ne assumo la responsabilità - e le selvagge aggressioni che esso ha subito. Potrei addirittura raccontare che talvolta è stata direttamente la mano pubblica a realizzare interventi che hanno stravolto l'assetto idrogeologico e che sono stati poi per larga parte responsabili di distruzioni e morti. A Sarno, nel bel mezzo del vallone Santa Lucia che normalmente sarebbe servito per canalizzare l'acqua piovana e i materiali che essa trascina con sé - sono visibili ancora oggi quattro manufatti. Non si tratta di opere abusive, onorevole collega relatore, ma addirittura di quattro opere pubbliche realizzate nel passato dall'ente locale: una scuola materna, una piscina comunale, un palazzetto dello sport e un centro sociale. Le colate laviche, prodotte dai distacchi della cosiddetta coltre piroclastica dalla montagna, scendendo a valle ed appesantendosi lungo il percorso di detriti, arbusti ed altro, trovando ostruito il vallone, deviavano il proprio corso verso l'edificato della frazione Episcopio, con una forza d'impatto dirompente: 137 morti nella sola città di Sarno. Una vera e propria ecatombe! In una situazione del genere come quella della Campania e di altre realtà, soprattutto nel Mezzogiorno, si può parlare di abusivismo di necessità? Certo, vi sono ricadute e drammi sociali inquietanti, ma vi è pur sempre la prioritaria ed indefettibile esigenza di tutelare la pubblica incolumità. Il discorso poi si impoverisce quando si pensi, com'è notorio, che questo provvedimento è dettato da un'esigenza manifestata durante l'ultima campagna elettorale Se per un verso è pensabile studiare un'iniziativa che, tenendo conto dell'emergenza abitativa, consenta alle pubbliche amministrazioni locali la realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare, come auspicato nella parte conclusiva dell'ordine del giorno di cui è primo firmatario il collega De Luca, (previa l'adozione - aggiungo - di particolari misure e di strumenti urbanistici adeguati) è per altro verso inconcepibile un generalizzato permissivismo. Ieri in Commissione ambiente è circolato un emendamento di cui già nei giorni scorsi si era avuta qualche anticipazione: una sorta di riapertura dei termini del condono del 2003, fissati nel dicembre 2004, che noi del Partito Democratico rigettiamo in modo assoluto e categorico. Sarebbe piuttosto auspicabile, signora Presidente, e concludo, un piano teso a restituire equilibrio e ordinato sviluppo al territorio, anche mediante la costruzione di nuovi alloggi, disciplinandone la fruizione e procedendo all'abbattimento di manufatti abusivi. Insomma, un intervento innovativo e salutare, ma rigoroso ed esemplare, in cui lo Stato reciti fino in fondo il proprio ruolo e per effetto del quale quella Regione, troppo spesso e talvolta ingiustificatamente identificata, ancora oggi in quest'Aula, come la terra delle vergogne, venga ricondotta a un'immagine differente a seguito del ripristino delle regole e del rispetto della legalità.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, devo anzitutto manifestare un certo disagio e imbarazzo perché negli interventi che ho ascoltato fino adesso sembra che il soggetto (quello che in qualche modo manifesta in tanti casi il bisogno) sia assente da questo dibattito. Si assiste a una rincorsa di quelle che sono state le inadempienze delle varie istituzioni - quella centrale e quella regionale e si perde di vista la realtà della situazione campana, come se si volesse rifare una ricostruzione storica - quasi dai tempi dei Borboni - di ciò che è accaduto e che accade. Dico subito che avrei voluto qualcosa di più estensivo, un decreto più utile e più opportuno. La considerazione di partenza è questa: se è vero, come il relatore ha affermato, che la possibilità dei campani di usufruire del condono 2003 avrebbe sanato gran parte (e quindi ben oltre il testo che ci viene proposto) la situazione attuale, allora vuol dire

È chiaro che all'interno di un abusivismo devastante nel nostro territorio andrebbe fatta una opportuna e doverosa differenziazione. È anche vero, per completezza, che il territorio campano è tutto vincolato:

federalismo, un funzionario di una qualsivoglia sovrintendenza possa sovrapporsi all'autorità di un Consiglio comunale eletto rispetto ad alcune iniziative. Proprio nel tempo in cui si delega ai territori, siamo in presenza di un centralismo che detta le condizioni. Non ho paura a dire ciò, perché non vorrei che questo dibattito risentisse di un'impostazione ideologica, secondo cui tutto quello che dalle nostre parti si fa è camorra, è malavita. Non è vero: ci sono tantissime persone che all'interno di loro pezzi di terra, lontano dalle zone a rischio

Anche oggi ci è toccato sentire il pistolotto rispetto all'emergenza della Campania. Ciò riguarda senz'altro un'aggressione, a mio avviso anche indiscriminata, perché ci sono sicuramente casi da contrastare e che tante volte non lo sono. Ma chi li deve contrastare? Quelle istituzioni che oggi sono inadempienti, che lo sono state. Chi deve vigilare?

si poteva procedere ad un'acquisizione coattiva in luogo delle demolizioni, vista anche l'emergenza abitativa della Campania; si poteva infine delegare la Regione affinché intervenisse nel merito della questione. A mio avviso, si è fatto poco, si è fatto poco, in quanto l'emergenza in maniera demagogica non verrà risolta, perché - lo hanno ricordato - gli abbattimenti sono oltre 60.000: anche economicamente è insopportabile mettere in pratica queste disposizioni. Allora, se è vero che una volta si ricorre alla politica e una volta alla scienza giuridica, dico che la Carta costituzionale è diritto ma è anche buon senso,

G101 affronta un argomento che secondo me comunque in Aula - e chiedo attenzione al Governo - è utile esaminare; certo non mi esimerò anche dall'intervenire nel dibattito che si è aperto, perché è un gioco di rimpalli. Capisco, senatore Villari, le aspettative - non solo le sue - politiche ma anche pratiche, probabilmente, di alcuni cittadini campani che volevano vedersi condonato l'abuso, però, davvero mi chiedo, politicamente e culturalmente, che messaggio stiamo mandando. Chi si costruisce una casa rispettando le norme, quindi chiedendo tutte le autorizzazioni (certo è complicato, certo la burocrazia è tanta) lo fa però seguendo appunto delle regole; chi invece costruisce la casa dalla sera alla mattina,

sia due volte devastante e pericoloso, non solo quindi da un punto di vista culturale del messaggio che si invia (le regole ci sono, però, certo, se poi qualcuno non le rispetta non importa, perché tanto poi arriverà un condono, o un decreto, o un condono-decreto, o ma è pericoloso anche da un punto di vista pratico, di quello che comporta un'abitazione abusiva in un territorio come quello campano, in particolar modo, per esempio, in quelle località dove vi è il rischio di un'eruzione vulcanica, dove vi è la possibilità che un vulcano si risvegli, in quanto poi bisogna anche evacuare un territorio. Dipende, certo, dalla portata dell'eruzione, dall'intensità, sicuramente avere delle costruzioni abusive che non rispettano alcun vincolo e che impedirebbero anche le vie di scorrimento e di evacuazione, credo sia una questione da prendere in considerazione, su cui porre l'attenzione prioritariamente,

L'ordine del giorno che abbiamo presentato, e su cui chiedo l'attenzione del Governo, si riferisce ad un ospedale che è stato costruito nel quartiere Ponticelli di Napoli. Non è un edificio abusivo: è stato costruito - immaginiamo - con tutti i permessi.

che dovrebbe essere uno dei più grandi dell'Italia meridionale - 4.050 posti di letto e 190 milioni stimati - si trova attualmente nella zona gialla, ossia in quella

10-12 chilometri è la zona rossa, oltre è la zona gialla: le zone sono state fatte seguendo i confini amministrativi. Di conseguenza, l'Ospedale del Mare si trova a 8 chilometri dal centro del vulcano; in altre parti la zona rossa si estende fino a 12

esistere una situazione del genere, in cui - ripeto - nella migliore delle ipotesi l'ospedale è da evacuare. Credo che l'occasione di questo decreto, che ritengo davvero devastante dal punto di vista politico

ho chiesto di intervenire in questa discussione generale dopo avere letto il testo di legge che la maggioranza ci propone. È la natura veramente singolare, quanto pericolosa, di questo decreto-legge che mi induce a prendere la parola per fare semplici ma - credo - doverose considerazioni. Sono lustri che le forze di centrodestra, con la Lega in testa - devo dirlo - lanciano vere e proprie invettive verso il Mezzogiorno, in particolare Le cause di giudizi duri, e non di rado offensivi, sono da ricercare nel modo con cui si amministrano quelle terre e nei comportamenti degli abitanti, non rispettosi delle regole, inclini a commettere illegalità e illeciti di ogni sorta e soprattutto alla ricerca di espedienti per raggirare la legge.

Non è vero che uno dei motivi ricorrenti della vostra propaganda è quella di ergervi a tutori delle leggi e della legalità denunciando che nel Paese non c'è certezza del diritto e della pena? È questo che voi denunziate costantemente? Insomma, credo che mai come in questo caso ci troviamo di fronte ad un intervento governativo diretto a neutralizzare il lavoro, difficile quanto incisivo, della magistratura. Badate, per chi non lo sapesse: effettuare indagini e quindi processi per violazioni edilizie, soprattutto in aree popolose come la Campania, è a dir poco arduo. Quando alla fine, tra mille difficoltà, una giustizia ansimante, che opera tra mille difficoltà, giunge a decretare una pena che è l'unica in questo settore ad essere incisiva e che può lanciare un segnale di segnale di prevenzione, ecco che si fa avanti un Governo amico che pone un ostacolo giuridico invalicabile. Si neutralizza l'applicazione della pena. Ma dove siete, senatori della Lega? Non capisco. Non era la Campania per voi quell'area che addirittura il Vesuvio avrebbe dovuto cancellare? Erano posizioni estreme, naturalmente, quanto offensive. Perché queste invettive? Perché in quella terra vi sarebbe stata sempre e comunque violazione delle regole. Adesso che abbiamo una magistratura che applica le leggi, a fatica, e che vuole attuarle, che vuole difendere il territorio e l'ambiente, voi chiudete gli occhi e, come gli struzzi, mettete la testa sotto la sabbia. Non vedete che state approvando, o state per approvare, un decreto-legge, una normativa fondata sull'illegalità, che è praticamente un elogio all'illegalità? Questo è il messaggio che uscirà da questo decreto-legge: in Campania in particolare, ma un po' ovunque in Italia, si faccia quel che si vuole perché tanto, comunque, interverrà sempre un Governo amico che neutralizzerà l'applicazione della legge.

desidero esprimere una preoccupazione forte per l'aria che si respira nel Paese in questi giorni. Un'aria di condono di condono edilizio, l'ennesimo, che rischia di essere ancora più devastante di quelli già impattanti e drammatici che il Governo Berlusconi ha varato ogni volta che si è trovato a governare il Paese. Ora, mentre svolgiamo questa discussione, è in corso la conferenza stampa del Presidente del Consiglio e del ministro Tremonti per illustrare la manovra, all'interno della quale, con il fantasioso nome di emersione delle case fantasma, in realtà è contenuto l'ennesimo condono edilizio. E questo provvedimento

pasticciato. Nella relazione che l'accompagna è scritto a chiare lettere che riguarderebbe circa 600 casi (le 600 abitazioni dell'isola di Ischia). Come è evidente - e come ha detto anche il relatore, senatore Orsi - in realtà, ciò che si affronta con il provvedimento è cosa ben diversa e riguarda un

nella relazione di accompagnamento del disegno di legge del Governo. Il pasticcio nasce dal fatto che si fa finta di voler affrontare un problema cosiddetto sociale per poi estendere il tutto a un condono generalizzato. L'ha detto prima di me il senatore Maritati ed io non posso che ripetere le sue argomentazioni: se c'è un problema sociale si deve affrontare con gli strumenti propri

che, a partire da Ischia stessa ma in tutta l'area del Vesuvio e in tutta l'area della Regione Campania, quegli abusi sono stati commessi in larghissima parte su

per evitarne la demolizione. È questo l'aspetto grave su cui si dovrebbe avere l'onestà intellettuale - mi rivolgo a tutta la maggioranza - di dire che non è un problema sociale.

un condono edilizio che non può che essere - lo dicevo prima - un regalo alle ecomafie, alla criminalità organizzata. Ciò di cui si discuterà non è

proporrete una vera e propria sanatoria edilizia. In questo senso vorrei sfidare la ministro Prestigiacomo, che ha fatto una conferenza stampa insieme all'Arma dei carabinieri e ad altre forze dell'ordine denunciando le illegalità e giurando e spergiurando che non vi saranno più condoni edilizi,

Credo che oggi, proponendo questo provvedimento per la Campania, voi stiate aprendo la strada ad una situazione che riguarderà tutto il territorio. Vorrei concludere rivolgendomi al relatore, senatore Orsi, che nel suo intervento ha voluto rimarcare la responsabilità della Regione Campania in tutta questa vicenda per le leggi che la Regione aveva varato ai tempi del condono edilizio e che poi sono state impugnate dalla Corte costituzionale, ribaltandone il ragionamento. Credo che

unica forse tra le Regioni meridionali, riuscì a fare un esercizio di politica seria di difesa del territorio cercando di restringere il condono edilizio fatto da Berlusconi nel 2003, che era stato uno scempio.

cercò di limitare al minimo gli scempi che quel condono edilizio di Berlusconi aveva compiuto in tutto il Paese.

sostanzialmente, da tutti i colleghi della Commissione ambiente e da gran parte dei colleghi campani del mio Gruppo. Noi abbiamo scelto di non presentare emendamenti a questo disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle demolizioni e di affidare la nostra posizione contraria - che verrà poi argomentata in sede di dichiarazione di voto dal senatore De Luca, ma che già molti colleghi hanno per vari aspetti illustrato - a a un ordine del giorno, che acquista tanto più valore dopo aver ascoltato la relazione del senatore Orsi. La relazione del senatore Orsi, molto precisa e molto puntuale nel ricostruire la successione degli eventi che, secondo lui e secondo la maggioranza, renderebbero necessario questo intervento legislativo, ha un limite vistoso dal mio punto di vista. Essa parla del fenomeno dell'abusivismo edilizio come se fosse qualcosa di completamente diverso da ciò che è, come se fosse un problema essenzialmente di disagio sociale. Del resto, abbiamo sentito anche gli interventi di alcuni colleghi, come ad esempio quello del senatore Villari, descrivere l'abusivismo come non si sentiva più fare da qualche decennio: come se fosse, nella gran parte dei casi, il problema di persone povere, semplici e diseredate che, lavorando di notte e di domenica, si costruiscono la propria casa. Naturalmente esistono anche casi di questo tipo, che vanno affrontati - anche questo è stato detto - con gli strumenti ordinari che sindaci, prefetti e Regioni hanno a disposizione nel caso in cui ordinanze sindacali o, come nel caso della Campania, ordinanze penali decidano la demolizione di immobili abusivi. Ma l'abusivismo edilizio è altro. Ed è drammatico constatare che la maggioranza nel 2010 ancora pensa a quello che è uno dei grandi mali del nostro Paese in termini assolutamente inadeguati a raccontarlo e, ancora di più, a fronteggiarlo.

agli aspetti legati alla difesa del paesaggio, ma l'abusivismo edilizio, prima di essere un problema di impatto sul paesaggio, è un problema di insicurezza per milioni di italiani che vivono in case costruite illegalmente dove case non si sarebbero dovute costruire. Nel nostro ordine del giorno noi forniamo anche alcuni dati che riguardano la Campania, ma che si potrebbero verificare del tutto fondati anche per molte altre Regioni italiane, in particolare per Regioni del Mezzogiorno. Abusivismo edilizio significa che, per esempio, in Campania non da quando ha governato il centrosinistra, colleghi della maggioranza, ma negli ultimi 30-40 anni, secondo i dati del CRESME (e non secondo dati di parte), tra un quinto e un terzo di tutte le nuove costruzioni è illegale. Ciò significa che queste costruzioni molto spesso sono realizzate dove - lo ripeto - non si sarebbe dovuto costruire: in aree a rischio sismico, a rischio vulcanico, a rischio idrogeologico. Gli ultimi decenni sono disseminati di tragedie che dimostrano come questo problema abbia provocato centinaia di vittime: dalla Calabria alla Sicilia, alla Campania. Vittime che hanno pagato un prezzo altissimo al fatto di vivere dove non dovrebbero esserci abitazioni. Questo è il problema dell'abusivismo edilizio. Il problema dell'abusivismo edilizio è un problema di legalità e di criminalità. A questo proposito cito un unico dato: due terzi di tutti i Comuni del Mezzogiorno che sono stati sciolti dal 1991 ad oggi (quindi sostanzialmente negli ultimi vent'anni) per infiltrazioni criminali sono stati sciolti per vicende che avevano a che fare anche con l'abusivismo edilizio. Altro che abusivismo di necessità! Parliamo di grandi speculazioni, di interi quartieri sorti illegalmente, in Campania ma non solo. Questo è il problema da prendere di petto, e continuare ad affrontarlo con norme che in qualche misura, in maniera più o meno estensiva, danno il segnale che prima o poi lo Stato arriva e se

che hanno preceduto e seguito gli ultimi condoni edilizi. Il senatore Ferrante ricordava che in queste ore il Governo sta annunciando al Paese la quarta sanatoria edilizia generalizzata. Io voglio ricordare che di queste quattro sanatorie, tre portano la firma di Governi Berlusconi, anzi portano la firma dell'accoppiata Berlusconi-Matteoli: quella del 1994, quella del 2003 e questa del 2010.

G100 (testo 2), su cui immagino che il parere del relatore e del Governo sarà contrario, anche perché nel dispositivo si impegna il Governo a non fare qualcosa che nel frattempo ha già fatto, cioè a non procedere a nuove e ulteriori sanatorie edilizie.

E noi a questa idea non ci rassegneremo mai: ci siamo battuti contro il condono del 1994, ci siamo battuti contro il condono del 2003, ci batteremo in Parlamento e nel Paese contro il terzo condono edilizio firmato Berlusconi. Per tale motivo ci battiamo anche contro questa norma apparentemente minore e che fortunatamente, anche per la nostra intransigenza, non è arrivata a riaprire i termini è arrivata a riaprire i termini del condono edilizio del 2003, ma che in ogni caso dà sempre lo stesso segnale: violate la legge che tanto prima o poi arriverà una norma che vi metterà in regola.

Signor Presidente, colleghi senatori, desidero innanzitutto ringraziare il relatore, senatore Orsi, che ha coerentemente riferito all'Aula il lavoro svolto in Commissione. Il relatore Orsi non ha solo puntualmente illustrato i motivi che hanno legittimato l'intervento del Governo, ma ha anche motivato le ragioni politiche e sociali che sottendono all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

invece, in alcune affermazioni fatte dal collega Villari: qui si tratta di restituire ai cittadini della Campania un diritto sacrosanto che è stato loro negato.

questione pregiudiziale che è stato violato un principio di uguaglianza, che esso è stato violato dalla Regione Campania che a suo tempo aveva deciso

noi siamo quelli del Governo che hanno l'ambizione di risolvere le questioni. Ricordo qui una frase di Bottai: siamo al Governo per fare la rivoluzione.

In Campania c'è un problema gravissimo, e i colleghi campani che sono presenti in Aula sanno bene che si tratta di abusi di necessità.

di aderire ad una legge dello Stato che introduceva il condono. Poi c'è tutta un'altra riflessione che dobbiamo fare e che deve fare

che non hanno mai proceduto a fare una pianificazione territoriale. Cosa facciamo in presenza di un'inerzia da parte delle Regioni? Dobbiamo affrontare e analizzare sottoscritto un emendamento - come ricordavano alcuni colleghi - che sosterrò,

quando si afferma che sarebbe impossibile stabilire l'epoca esatta della costruzione del manufatto abusivo. Ci sono le aerofotogrammetrie, le mappe catastali, i rilievi fotografici, altri documenti concernenti i lavori, come le fatture, e tante altre documentazioni che si possono produrre. Penso che

debba indirizzarsi verso l'approvazione di questo provvedimento.

del quale, in sede di replica, devo necessariamente dare conto di qualche intervento ed anche confutare alcune delle affermazioni che ho ascoltato. Nel paradosso di questo dibattito vi è la contestazione dei dati proposti dal relatore sul numero degli abusi: faccio presente che questi dati sono contenuti in un ordine del giorno sottoscritto dai senatori di maggioranza e sono il frutto del rapporto di Legambiente dell'anno scorso e di una dichiarazione del capo della procura della Repubblica di Napoli. Dico questo

che annuncia una sorta di conflitto di attribuzione, perché andremmo ad intervenire su sentenze passate in giudicato, non sta in piedi per due ragioni: in primo luogo perché

un'osservazione nei confronti della Corte costituzionale che, piaccia o no, colleghi Andria e Ferrante, ha dichiarato illegittime le leggi della Regione Campania. In questa sede, se vogliamo ragionare su un equilibrato rapporto tra le funzioni dello Stato, non possiamo esaltare una legge che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, quindi non appartenente all'ordinamento giuridico ed alla basilarità dei diritti dettati dalla nostra Costituzione. Ricordiamo questa affermazione per il futuro.

numerosissime Regioni, molte delle quali amministrate dal centrosinistra (Toscana, Emilia-Romagna, Basilicata), hanno legiferato in tema di condono, e lo hanno fatto nel rispetto dell'ordinamento, ed hanno interpretato nel loro territorio l'applicazione del condono anche con criteri rigorosi e restrittivi come hanno fatto molte Regioni governate dal centrodestra, compresa la Regione Liguria, della quale all'epoca ero l'assessore regionale competente. Se la Regione Campania non è stata in grado di fare una legge nei tempi stabiliti dalla Corte costituzionale e nella legittimità dell'ordinamento garantito dalla Corte Costituzionale, la Regione Campania ha sbagliato, e questo errore è uno dei presupposti della situazione di emergenza. Non credo che sia ragionevole l'affermazione fatta dalla collega Mazzuconi, che ha ricondotto alcune delle nostre affermazioni fatte nel dibattito ad una generica critica nei confronti del Sud, perché sulla materia del condono e dell'abusivismo edilizio la Regione Campania si è distinta per inefficienze ed incapacità rispetto alle altre Regioni del Sud, che hanno legiferato e tentato di governare il fenomeno, tanto è vero che oggi interveniamo sulla situazione di emergenza della Regione Campania che non è diffusa a tutte le aree che con la Regione Campania possono condividere alcune problematiche di fondo. le critiche (che lei ha definito al limite dell'insulto) che ha trovato nelle mie parole nei confronti delle amministrazioni della Regione Campania sono inferiori alle affermazioni che lei ha fatto citando alcuni casi specifici di incapacità di governo del territorio di quella Regione.

per esercitare le proprie competenze. *(Applausi dal Gruppo* *PdL)*. Credo che sia inaccettabile richiamare la responsabilità dell'assenza di un piano di intervento della Regione Campania, collega Mazzuconi, perché le ricordo che la Giunta si è insediata 12 giorni fa e avrà sei mesi di tempo

concede il tempo strettamente necessario alla Regione Campania per riappropriarsi del governo del territorio e delle relative conseguenze anche dal punto di vista della gestione dell'emergenza abitativa che - mi rivolgo ancora al collega Andria - non è responsabilità dello Stato: lo Stato di queste cose non si occupa in nessuna Regione, collega Andria. Di questi temi si occupano le Regioni e le Province. Se la Regione Campania non è stata in grado di gestirli, non credo che possiamo richiamare la responsabilità dello Stato, per la costrizione, che oggi ci vede tutti a celebrare un fallimento, che impone al Parlamento di intervenire perché bisogna risolvere un problema che il decennio di Bassolino non è stato in grado di gestire sul territorio.

Se dovessimo chiedere ai senatori presenti in Aula chi è favorevole all'abusivismo, sono convinto che nessuno alzerebbe la mano. Però qui stiamo parlando di una Regione d'Italia, la Campania, dove un procuratore ha scelto di procedere, secondo le leggi vigenti, all'abbattimento di alcuni manufatti.

Ho ascoltato con molta attenzione nei giorni scorsi il dibattito in Commissione. Ringrazio il presidente D'Alì per il grande impegno profuso

il principio di non discriminazione non permette di discriminare la Regione Campania nei confronti di tutte le altre Regioni che nell'anno 2003 hanno potuto usufruire di una legge nazionale. alla quale mi pare che buona parte dei colleghi guardino con una certa deferenza, ha reso illegittima. Ciò sta allora a significare che una parte del popolo italiano non ha potuto usufruire di leggi nazionali che in quel momento vigevano e non ha potuto trarre i vantaggi o gli svantaggi necessari inerenti alla legge stessa.

stiamo parlando di un provvedimento temporaneo, fissato nel tempo, che riguarda un certo tipo di casa, ovvero la prima casa di abitazione per coloro che la abitano stabilmente. per coloro che la abitano stabilmente. Ciò sta a significare che i provvedimenti di demolizione potranno andare avanti per tutti gli altri abusi in Campania

Aggiungo, come Sottosegretario delegato alla casa, che è in corso da parte del Governo l'approntamento del piano casa, che potrebbe anche dare una mano in questo senso. Senatore Molinari, non riapriamo i termini.

da due anni sto aspettando ancora una risposta dal Notariato italiano. Probabilmente questo Paese ha bisogno, da parte di tutti e non solo del Governo, di elementi strutturalmente più forti sul piano della legalità. Senatore Ferrante, e mi rivolgo anche al senatore Russo, che parla di responsabilità anche di amministratori di centrosinistra, di centrosinistra, se la Campania nel 2003 scelse di restringere gli scempi del condono Berlusconi, mi dica lei che risultato abbiamo ottenuto dal 2003 ad oggi. di restringere gli scempi del condono Berlusconi, oggi forse dovremmo parlare di qualcosa di diverso. Invece, purtroppo, stiamo parlando della Campania che non ha potuto beneficiare delle leggi nazionali e che quindi fa riferimento ancora al condono dell'anno 1994. Concludo. Senatore Andria, lei è stato presidente di una importante Provincia italiana.

le opere pubbliche non le costruisce il Governo in modo abusivo o su terreni che sul piano idrogeologico non presentano la necessaria sicurezza. la necessaria sicurezza. Ascrivere al Governo responsabilità che non ha credo sia improprio; tutti insieme dobbiamo provvedere ad ascrivere le responsabilità agli amministratori locali.

sciolto per condizionamenti camorristici, l'Arma dei carabinieri ha posto sotto sequestro 74 palazzi abusivi, oltre 500 appartamenti. Di questi palazzi ne sono già stati demoliti la maggior parte, grazie all'azione di pressione esercitata anche da questa prefettura in nome del Governo, ed alla collaborazione della Commissione straordinaria che ha operato in quel Comune fino al novembre scorso». Non abbiamo quindi interrotto nessuna demolizione in questi tre anni. Si tratta però oggi di un provvedimento di carattere urgente sul tema della prima casa, al quale pregherei pertanto di riservare la debita attenzione. Chiudo rivolgendomi ai senatori dell'opposizione, che naturalmente hanno espresso le loro perplessità, ricordando loro

che prevedono l'obbligo di stendere i piani di governo del territorio, perché questo è quello che manca in Campania. Oggi le isole sono tutte coperte da un vincolo assoluto,

che preveda eventualmente, se lo riterrete, anche lo scioglimento dei consigli comunali non solo per ragioni legate alla criminalità organizzata, ma forse anche per eccesso di abusivismo nei territori.

per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.2 e 1.3, sulle quali il parere è di contrarietà semplice». parere è di contrarietà semplice». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.100 (testo 2), 1.350 e 1.700, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo

di riformulazione, però è chiaro che addirittura si coinvolge la necessità di grande attenzione anche da parte di una delle più grosse Regioni italiane, con la speranza che poi, come spesso accade, ci si ricordi subito dopo l'adozione di questo ordine del giorno di quello che ci si è impegnati a fare e non a un anno dall'adozione dello stesso, quando magari si deve affrontare un'altra emergenza.

della lettera inviata il 22 maggio scorso dal Presidente della Repubblica, con la quale il Capo dello Stato ha ricordato "i criteri per l'adozione dei decreti-legge ed i caratteri di omogeneità che ne devono contrassegnare i contenuti", anche con specifico riferimento alle prerogative costituzionali attribuite al Presidente della Repubblica. Pertanto, la Presidenza, dando seguito alle puntuali indicazioni sopra richiamate, ha attentamente valutato l'attinenza degli emendamenti al testo del decreto‑legge in esame, il cui contenuto è limitato alla sospensione delle demolizioni - disposte a seguito di sentenza penale - di immobili siti nella Regione Campania, destinati a prima abitazione. Sono dunque improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.2 e 1.3, del senatore Nespoli, concernenti riapertura di termini per condono edilizio e sanatoria di abusi edilizi in Campania; 1.100 (testo 2), del relatore, su finanziamento interventi piano straordinario edilizia residenziale e 1.0.2, della Commissione, concernente valorizzazione alternativa di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 1.100a, della senatrice Vicari, recante norme in materia di subcontratto di fornitura; 1.0.1 (testo 2), della Commissione, concernente cause di sospensione di processi.

sull'andamento dei lavori. Rispettiamo le indicazioni della Presidenza, soprattutto in conseguenza dell'intervento del Presidente della Repubblica, però, io credo che quest'Aula e il Governo si debbano rendere conto che questo decreto è un piccolo palliativo rispetto alla problematica che affrontiamo, così come emersa anche dal dibattito svolto in quest'Aula. Ritengo che, con i tempi che questo provvedimento dà alla Campania, ci sia poi la necessità, in questo arco temporale, di provvedere ad incidere, rispetto alla questione posta, con una norma legislativa che dia le risposte doverose in termini di parità di trattamento dei diritti ai cittadini campani, rispetto non solo al condono del 2003, ma anche all'applicazione della legge del cosiddetto piano casa che la Regione Campania ha approvato alla fine del 2009. Ad ogni modo, ribadisco il ritiro dell'emendamento

gli effetti della sospensione delle demolizioni degli immobili abusivi, includendo nel provvedimento di sospensione anche gli abusi commessi in aree vincolate. Con questo emendamento del relatore si prevede che, nel caso degli abusi compiuti in aree vincolate, la sospensione non abbia la durata di più di un anno, cioè non duri fino al giugno 2011, ma abbia fine il 31 dicembre 2010, ma resta un principio molto grave, ossia quello di ammettere in qualche modo in questo caso dilatorio di provvedimenti penali passati in giudicato abusi compiuti in area vincolata. Inoltre, il riferimento alla futura redazione del piano paesaggistico lo trovo davvero surreale, perché capovolge l'ordine che dovrebbe esserci tra sviluppo urbanistico e pianificazione paesaggistica. Noi stiamo parlando di abusi che dovrebbero essere stati commessi entro il 2003, quindi i vincoli con cui questi abusi dovrebbero fare i conti sono quelli allora vigenti. In questo caso, invece di prevedere, come dovrebbe essere la norma, che lo sviluppo urbanistico si adegui alla pianificazione paesaggistica, si prevede il contrario, cioè si prevede che sia la pianificazione paesaggistica ad adeguarsi allo sviluppo urbanistico di fatto. È evidente - non credo sia una previsione azzardata - che la Regione Campania, nel redigere - ammesso che lo rediga in tempo utile - il suo piano paesaggistico, lo ritaglierà sullo sviluppo urbanistico di fatto che c'è stato, quindi per esempio farà in modo che le aree a più alta densità di abusi edilizi non siano ricomprese tra quelle su cui vige un vincolo assoluto di inedificabilità. Quindi credo che l'emendamento in esame introduca un precedente assolutamente

decreto-legge, che reca la temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania, non risolve sicuramente il problema, ma si limita a posticiparlo nel tempo. Si prevede solo un rinvio e non si dà, quindi, una soluzione adeguata per contemperare quelli che sono degli interessi contrapposti: da un lato, la tutela al diritto all'abitazione e, dall'altro, la salvaguardia la promozione della legalità e la difesa di un territorio già così fortemente provato da un abusivismo di cui, spesso, si sono dovute tristemente interessare anche le cronache, per le conseguenze mortali e gli scempi paesaggistici. paesaggistici. Vorrei ricordare a tutti voi che da un terzo a un quinto delle case costruite in Campania negli ultimi decenni è illegale, e non di rado in tutto questo viene coinvolta la criminalità organizzata. I Comuni a grave rischio idrogeologico sarebbero circa l'80 per cento La Campania ha una percentuale del 17 per cento del territorio esposto a rischio frane e alluvioni e negli ultimi anni questo dato si è palesato in più occasioni in tragici eventi. Un provvedimento opportuno avrebbe dovuto contemplare quello che è un effettivo programma che potesse valutare caso per caso l'effettiva necessità della violazione e, casomai, prevedere misure a favore di quegli individui sprovvisti di alloggio, come donne con bambini, anziani e non ultimi i diversamente abili, attraverso quelli che sono dei concreti programmi di edilizia pubblica volti al loro riallocamento. Al contrario, non si è fatto nulla e non si fa nulla in questo disegno di legge. Si procede piuttosto, come al solito, con una sanatoria occulta, mentre nessuna politica viene proposta per risolvere l'emergenza abitativa che investe indubbiamente una Regione popolosa come la Campania. una normativa, al contrario, che permettesse di abbattere veri e propri scempi che deturpano il paesaggio e spesso e volentieri mettono a rischio vite umane, in quanto costruiti su terreni non sicuri, arroccati su montagne a rischio di smottamento, ma, nello stesso tempo, sarebbe stato altrettanto urgente affiancare a questi programmi di demolizione idonee politiche abitative come prima sollecitavo. Quindi, noi invitiamo a riflettere ancora su questa temporanea sospensione. Diventa sempre più improrogabile una presa di posizione forte e determinata, soprattutto nei confronti di quelle che sono le costruzioni abusive. Il problema andrebbe risolto a monte, bloccando sul nascere con controlli a tappeto, più serrati, duri e che non facciano sconti a nessuno. Solo un braccio di ferro in tal senso, quindi all'origine del fatto stesso, avrebbe evitato di giungere indubbiamente a questo punto e di adottare inappropriate soluzioni temporanee. Naturalmente non siamo d'accordo, nello

di risolvere la questione in altro modo. La Campania, però, crediamo non abbia bisogno di provvedimenti tampone, ma di un insieme di politiche serie. Tra l'altro, devo dire che

che riguarda proprio i processi in atto. Vi invito a farceli capire, perché oggettivamente non se ne capisce il senso. Per queste ragioni, dal momento che il provvedimento non offre alcuna soluzione in tal senso, anzi ha se possibile, ulteriormente peggiorato nel passaggio, come ho detto, in Commissione, dichiaro il voto contrario del mio Gruppo.

amministrativo e urbanistico creato dalla Regione Campania. Ciò non fa altro che evidenziare come Paese Italia sia formato da più Paesi. Allora, ben venga il federalismo che il nostro partito proclama da 25 anni. Questa Regione rossa ha tentato, con un provvedimento che andava contro ogni logica,

irrazionale, rendendo il territorio pericoloso anche per i suoi abitanti. Gli studenti di urbanistica

Già in quell'anno si erano create delle situazioni nella città di Napoli - allora per problemi sanitari

rispetto alle quali ci sentiamo fortemente responsabili. Mi spiace invece che molti colleghi che abitano in quella Regione, ma che siedono nella parte sinistra dell'Aula, non abbiamo avuto il coraggio di dichiarare queste cose.

Io non mi meraviglio di nulla di ciò che viene presentato dal Governo, non mi meraviglio delle cosiddette case fantasma, vale a dire due milioni di case abusive che verranno sanate con la manovra

perché evidentemente bisogna rispondere al pagamento di una cambiale elettorale che il centrodestra aveva promesso nelle scorse elezioni regionali e che oggi mette all'incasso,

ricordare anche al sottosegretario Mantovani che il Presidente della Repubblica, con lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 2009, in occasione dell'esame del decreto-legge sul cosiddetto caso Englaro, ha avuto modo di rilevare come «il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente al legislatore di disattendere la soluzione che - nel caso di specie - sia stata già individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall'ordinamento giuridico È infatti principio consolidato in tutti gli ordinamenti democratici che la legge sopravvenuta non possa e non debba influire sul diritto sul quale il magistrato si è già pronunciato con un provvedimento passato in giudicato: così come il giudice non può sovrapporsi alla legge, attribuendo o negando beni giuridici che l'ordinamento non consente di attribuire o di negare». Pertanto, non è concepibile ciò che questo decreto-legge pone in essere. D'altra parte, vorrei ricordare a me stesso, ma non sfuggirà e non sfugge né al Governo, né al relatore, né ai colleghi, che la demolizione è una sanzione accessoria della sentenza di condanna penale, per cui siamo di fronte ad una condanna penale che ha che ha portato l'autore del reato ad essere condannato e, come sanzione accessoria, ad essere obbligato a demolire. Ecco perché l'intervento del Governo appare del tutto inopportuno.

certamente alcuni. E dunque, chiedo al relatore, al Governo e ai colleghi chi deve verificare, chi deve fare la ricognizione della situazione. Non vi è una situazione fotografata. Di fatto, è un condono chiaro e puntuale perché non sappiamo quali sono i soggetti. Tra l'altro, vorrei ricordare che l'articolo 34 della legge sul condono prevede che possono comunque avere i benefici del condono (nel caso di specie anche della sospensione, perché dovrebbe essere estesa)

Il decreto-legge che voi vi accingete ad approvare non parla di tutto ciò. Di tutti i problemi che la casistica porrà, questo decreto-legge non parla, lasciando volutamente nella nella nebbia tutti i vari casi che si andranno configurando. Noi come Italia dei Valori riteniamo che questo sia un provvedimento ingiusto sia un provvedimento ingiusto e che, tra l'altro, esso differenzi posizioni giuridiche uguali, perché ci sono soggetti che hanno già subìto la demolizione

pedagogicamente, nei confronti dell'intero Paese, e non solo dei cittadini della Campania, è quanto di più sbagliato il Governo potesse proporre. Presidente, onorevoli colleghi, io credo che di questo decreto, probabilmente, sfugga il contesto.

Ma qual è il contesto della richiesta di questo decreto per la Regione Campania caro sottosegretario Mantovani? Esso è legato a un provvedimento del magistrato qualche modo, finisce per inglobare tutto rispetto ad una situazione che da decenni vive una propria illegalità;

Noi dobbiamo ragionare su questo contesto e mi dispiace che il senatore Leoni, probabilmente tradendosi, voluto far riferimento a un provvedimento adottato nel 2003 dalla Regione Campania per tentare di ridurre il fenomeno grave dell'abusivismo nella Campania rispetto a un condono del livello nazionale. Altro che dileggio nei confronti della Corte costituzionale! La questione è un'altra è la stessa motivazione addotta dal senatore Orsi, caro senatore Monti, quando, forse tradendosi, ha fatto riferimento alla vicenda dei rifiuti. È la logica

Mi sembra veramente un atteggiamento irresponsabile che l'Aula del Senato non si può permettere in una situazione come questa. Tra l'altro, nel momento in cui si definisce un provvedimento del Governo che cerca di reperire 2 milioni di case abbandonate, c'è una logica oramai perversa, un atteggiamento incline al condono, che abbassa il livello di legalità.

quando in quell'occasione si tentò di frenare quel condono del 2003, la Regione Campania faceva riferimento proprio ad un senso di maggiore responsabilità, anche essendoci una responsabilità da parte degli amministratori,

L'amarezza di questo dibattito, lo dico da campano, è quando ci si vuol nascondere dietro ad un'emergenza sociale tragica

in questo decreto abbiamo tentato di dare un contributo, anche con qualche risultato positivo: cosicché, non è un ennesimo condono. Non è solo il richiamo del Presidente della Repubblica, ma è il modo in cui il Governo del Paese si fa carico di una visione più ampia. Si è fatto riferimento alla provincia di Salerno, alla provincia di Salerno, che ha confiscato beni e ha abbattuto abusi, e rispetto a questa condizione non facciamo riferimento alla Corte costituzionale, per l'amor di Dio,

quando la Regione Campania ha prodotto una legge rispetto alla provincializzazione dei rifiuti, il Governo l'ha impugnata, per produrre il decreto-legge n. 195 del 2009 sui rifiuti, che fa riferimento alla provincializzazione. Insomma, cerchiamo di smetterla: lo dico con grande senso di preoccupazione e di responsabilità.

anche rispetto ad un piano di edilizia popolare e tramite un raccordo con gli enti locali. Non si tratta di sospendere le demolizioni e restare fermi, perché fra sei mesi non potremo affidarci alla fatalità o allo Spirito Santo. La questione resterà lì.

Un Governo che guarda agli interessi generali del Paese non solo rispetta un provvedimento di un organo autonomo come la magistratura, ma tenta di dare una risposta non rinviando il problema,

al confronto, ma sul piano di un proposta complessiva che salvaguardi questo principio di legalità e cerchi di finirla con la logica dell'abusivismo, perché non possiamo vivere di tentativi disperati, disperati, a fronte di una situazione tragica. Probabilmente l'unico motivo di disperazione rispetto al panorama che viviamo è un decadimento della rappresentanza ed uno svuotamento delle istituzioni: con la logica del delegare ad altri e ai vari commissari

a parte i colleghi che hanno vissuto il dibattito in Commissione, ho avuto l'impressione che vi siano delle lacune conoscitive rispetto sia alla relazione sia al testo del decreto.

una definitiva eliminazione delle demolizioni, peraltro prescritte dalla magistratura. Bene ha fatto il relatore, nelle cui considerazioni interamente mi ritrovo, ad assimilarlo alla proroga degli sfratti. Qui c'è un'esigenza assolutamente chiara, netta e socialmente rilevante che è stata segnalata al Governo dalla magistratura in prima battuta - come ha ricordato il il sottosegretario Mantovani - per la mole enorme delle incombenze che dovrebbero derivare dall'esecuzione delle sentenze di demolizione (e qui parliamo solo di demolizione e nulla osta che si proceda anche sul piano delle confische). È stata sollecitata soprattutto dai sindaci, la stragrande maggioranza dei quali rappresentata da una folta delegazione intervenuta in Senato

Quindi, è un provvedimento che non esaurisce la tematica, ma che pone le condizioni perché quando questa tematica verrà risolta, attraverso le proposte che farà il Parlamento e la stessa Regione,

in questa sede lo abbiamo completato con un differimento di sei mesi, ed ha un preciso e diretto riferimento assumendo la veste per la prima volta di importante strumento di *moral suasion* nei confronti delle amministrazioni locali, in questo caso della Regione, che devono provvedere alla redazione dei piani paesaggistici. Quindi, è un provvedimento che si pone in termini positivi nei confronti delle autonomie e degli enti locali, stimolandoli ad intervenire perché essi sanno che, qualora non dovessero adempiere a quanto gli viene richiesto perché si possa effettivamente avere un quadro complessivo della situazione, si ritroveranno con la situazione di oggi, forse ancor più aggravata. non tanto nel merito, quanto nella prudenza di una situazione che richiede un momento di pausa perché possa essere programmato un vero intervento che metta che metta i Comuni della Campania nella condizione di poter arginare il fenomeno gravissimo del disagio abitativo. C'è stato paradossalmente contestato il fatto che è un provvedimento che riguarda solamente la prima abitazione. Allora, si voleva un provvedimento che riguardava tutto l'abuso edilizio complessivo nella Regione Campania? È un provvedimento mirato; ha una problematica sociale che, riconoscendomi - ripeto - in tutto quello che ha detto il relatore Orsi - trova radici in altri tempi, in altri momenti, ma non voglio ritornare più di tanto sull'argomento.

derivanti proprio dall'esistenza di quegli edifici. Come si fa a dire pertanto che il Governo non è attento ai problemi della sicurezza quando, pur in presenza del disagio abitativo,

a prescrivere anche una revisione dei piani regolatori esistenti. Purtroppo, è stato dimostrato che molte delle disgrazie dovute a causa di dissesto idrogeologico sono avvenute in situazioni di piani regolatori approvati,

e scolastici che sono stati fatti dalla mano pubblica attraverso l'approvazione di piani regolatori, quindi in regime di perfetta legittimità, in zone di assoluto rischio e pericolo.

dietro qualcosa. Pur di andare contro l'ipotesi governativa è stato detto che il Governo si nasconde dietro la sentenza della Corte costituzionale: si dovrebbero nascondere, ma per la vergogna, dietro la sentenza coloro che l'hanno provocata, perché hanno privato una Regione di una possibilità di sistemazione del comparto edilizio in coerenza con quello che è stato fatto in altre parti del territorio nazionale.

il senatore De Luca non può certo realizzarsi attraverso uno scenario quasi post bellico di circa 60.000 demolizioni che dovrebbero essere fatte nei prossimi mesi, ammesso che la magistratura e gli enti locali abbiano le risorse necessari. Chi ha amministrato un ente locale sa benissimo quali sono gli oneri che incombono su un ente locale nel momento in cui si procede a un numero elevatissimo di demolizioni, dovendo pure provvedere al disagio abitativo e, quindi, a reperire alloggi e strutture per poter allocare le famiglie costrette ad abbandonare gli immobili destinati all'immediata demolizione. che dovremo tornare sull'argomento; per questo ci torneremo anche con iniziative legislative parlamentari; è per questo che la 13a Commissione del Senato dovrà affrontare questo argomento, prima che venga affrontato su altri fronti, d'intesa con la Regione Campania, che è la titolare della materia, per risolvere un problema che non è, ripeto, di denegata legittimità, è un problema serio dal punto di vista sociale, sul quale oggi si interviene con una prudenzialissima mossa di sospensione di appena un anno cosa significa un anno per le nostre amministrazioni - e di sei mesi per quanto riguarda la redazione dei piani paesaggistici. È una norma di saggezza e prudenza, che deve essere però accompagnata con senso di responsabilità dal nostro successivo intervento, dall'intervento della Regione Campania, dall'intervento degli enti locali che non possono ogni volta attendere l'opera

tutti coloro che hanno partecipato a questo dibattito. In Commissione, soprattutto, si è avuto un dibattito responsabile, ma trovo naturalmente su fronti assolutamente opposti la maggioranza

concretamente utile, per poter innescare un dibattito di carattere generale che non ha niente a che vedere con la situazione che stiamo affrontando e cercando di risolvere con senso di responsabilità e concretezza.

e purtroppo io, come tutti quanti voi, sono nominato con questo sistema elettorale, non sono un eletto. Siamo sempre più distanti dalla gente e non riusciamo a capire i problemi che ci sono in alcuni territori.

senatore Pedica. PRESIDENTE. Colleghi, chi vuole uscire esca, ma faccia terminare la seduta e soprattutto in questo momento faccia svolgere l'intervento al senatore Pedica. Grazie, signor Presidente,

organizzata dalla Polizia penitenziaria. Il numero dei detenuti ha raggiunto la cifra record di 67.542, a fronte di una capienza di circa 44.000 posti detentivi. Mancano 6.500 agenti di Polizia penitenziaria. Gli agenti sono costretti a fare turni di 8-9 ore senza che venga corrisposto uno straordinario. Coloro che vengono inviati in servizio di missione debbono anticipare i soldi. Un agente di Polizia penitenziaria è costretto a sorvegliare fino 150 detenuti, molti dei quali affetti da patologie infettive.

il Governo ancora oggi parla di assunzioni di 2.000 agenti, che non arrivano, e l'organico appunto è sottodimensionato; mancano 6.500 agenti non i 2.000, che vuole offrire

e che implodono, e lo stanziamento di risorse per il rinnovo contrattuale e il riordino delle carriere e la previdenza complementare. Non c'è ad oggi un ordine del giorno